L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. Comunico che, in data 29 marzo 2023, è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n.16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina»

recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi oggi, ha ridefinito il calendario dei lavori dell'Assemblea, che sarà comunicato domani, alle ore 14.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

Signor Presidente, il 15 giugno 2022 l'associazione Animal equality ha presentato alla Commissione europea una denuncia, per segnalare con forza gli abusi a danno dei polli da carne a rapido accrescimento, i cosiddetti polli *broiler*. Precedentemente l'associazione aveva presentato anche una petizione per chiedere di porre fine all'allevamento di questi animali, frutto di una selezione genetica, che crescono troppo in fretta e che sviluppano eccessivamente petto e cosce, le parti più vendibili sul mercato. Il loro organismo, dunque, non è in grado di sorreggere il peso innaturale raggiunto, con conseguenti problemi ai muscoli, agli arti, alle vie respiratorie e al cuore, determinando non solo problemi cardiocircolatori, ma anche ascite, dermatiti e serie difficoltà nel raggiungere acqua

raggiungono il doppio del peso, 2,5 chili. Sappiamo che l'unico obiettivo di questa selezione artificiale è quello di ottimizzare la produzione industriale di uno degli animali più allevati, sfruttati e macellati al mondo. I polli uccisi ogni anno per l'alimentazione umana, infatti, sono oltre 60 miliardi. Queste pratiche di allevamento sono palesemente in contrasto con l'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che riconosce gli animali come esseri senzienti, e con la direttiva n. 58 del 1998 sulla protezione degli animali negli allevamenti, che prescrive in particolare che agli animali non siano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili. Per questo ho presentato un'interrogazione in 9a Commissione, sottoscritta da molti colleghi. Siamo di fronte a veri e propri soprusi genetici: una realtà che riguarda altre specie, come, ad esempio, i maiali Duroc e i tori Blu belga, che sviluppano una muscolatura esagerata e deforme. Questa mutazione - chiamata doppia muscolatura - ha un unico intento: avere maggiore carne destinata alla vendita per massimizzarne i guadagni. Tutto questo non può essere ignorato. La legge n. 189 del 2004, che ha introdotto nel codice penale i delitti contro il sentimento per gli animali, è stata approvata proprio per arrestare le pratiche di maltrattamento. Contenuti, questi, che sono diventati principi costituzionali grazie alla nostra proposta, quindi, grazie al MoVimento 5 Stelle, che ha avanzato questo concetto culminato con la pubblicazione della legge costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022. Grazie alla nostra iniziativa, infatti, all'articolo 9 della Costituzione è esplicitato - nero su bianco - che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Considerata la crescente sensibilità dei cittadini italiani a riconoscere gli animali come esseri senzienti, dunque, è nostro dovere politico impegnarci affinché simili sofferenze non siano più causate né in modo diretto né in modo indiretto. Il dio denaro non può e non deve dominare.